«Roma 29 gennaio 2022 Cara Presidente, ho l'onore di comunicarLe, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 87 del 1953, che la Corte costituzionale, oggi riunita nella sua sede del Palazzo della Consulta, mi ha eletto Presidente. Firmato Giuliano Amato». In data 27 gennaio 2022, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del turismo, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e della cultura:* «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da

Signor Presidente, colleghi, nonostante procura generale della Corte dei conti e procura di Roma stiano indagando sull'approvazione postuma del CIPES, dopo la proposta dei ministri Giovannini e Franco del piano su Autostrade, malgrado il parere contrario della stessa Corte e dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nei giorni scorsi lo stesso CIPES, presieduto dal presidente Draghi, ha dato il via libera a un'operazione a perdere, con lo Stato che ci rimette circa 8 miliardi di euro regalati ai Benetton, quegli stessi signori dei caselli che hanno gestito le autostrade italiane, la gallina dalle uova d'oro, incassando ricchissimi dividendi senza fare manutenzione, causando la tragedia del ponte Morandi con 43 morti. "Il Tesoro ha telefonato": le pressioni del Ministro dell'economia per spianare Autostrade ai soliti fondi. Una fonte rivela al settimanale TPI le pressioni del Ministero dell'economia per favorire l'operazione CDP Atlantia: "Funzionari ministeriali telefonavano per invitare gli interessati a farsi da parte". Titolo del 12 novembre 2021. Su questa operazione, che ha registrato documenti mancanti, con potenziali concorrenti a cui non sono mai state fornite informazioni indispensabili, una *data room* aperta e poi improvvisamente chiusa, pressioni del Tesoro - come ha scritto Laura Maragnani su TPI - addirittura, per scoraggiare i possibili acquirenti in un'«opaca operazione» che lo Stato sta conducendo per acquisire Autostrade per l'Italia (Aspi), ho presentato numerose interrogazioni. Un'operazione che gira intorno all'88,6 per cento delle quote in mano ad Atlantia, la società in cui la famiglia Benetton fa la parte del leone, acquirente il consorzio HRA, composto da Cassa depositi e prestiti (51 dai fondi Blackstone e Macquarie, al prezzo di 21,3 miliardi di euro, contro i 13,8 miliardi che sarebbe costata la revoca della concessione. Come sono stati scelti i fondi *partner* dell'operazione, l'americano Blackstone e l'australiano Macquarie (tra i cui *advisor* c'è Claudio Costamagna,

Gli azionisti principali di Blackstone sono Vanguard Group e BlackRock, e sempre loro sono i maggiori azionisti del fondo Macquarie. In altre parole, Vanguard Group e BlackRock escono dalla finestra con la mega liquidazione di Atlantia e rientrano dalla porta con il nuovo consorzio, mentre Aspi, società strategica per l'Italia, viene controllata da fondi stranieri.